e, su iniziativa del presidente Ortega, sono già stati arrestati alcuni dei candidati presidenziali a lui concorrenti. Credo che dovremmo, nei modi e nelle forme che il Governo riterrà utili, elevare una vibrata protesta e che l'Europa debba assumere un'iniziativa. Ormai si stanno ripetendo nel mondo fenomeni assai preoccupanti. È di queste ore l'inasprimento della repressione in Birmania, la situazione del Venezuela continua ad essere una sorta di emergenza umanitaria e oggi il Nicaragua si aggiunge drammaticamente a questo elenco di disastri mondiali. Esprimendo solidarietà ai cittadini del Nicaragua, alle donne, agli uomini e ai giovani impegnati nelle proteste, duramente repressi e incarcerati, vorrei dire che l'Italia, per le tradizioni nobili di attaccamento ai valori di libertà e democrazia,

trasferirò la sua doverosa richiesta alla Presidente del Senato e intanto mi associo al cordoglio.

Signor Presidente, avendo ricevuto e acquisito il parere sugli emendamenti del relatore da parte del Presidente della Commissione bilancio, dato per favorevole il parere del relatore su un suo stesso emendamento, direi che il Governo avrebbe bisogno, dal momento che si tratta di un provvedimento congiunto che prevede sia le competenze del Ministero dell'interno che del Ministero della giustizia, una ragionevole sospensione di dieci minuti per poter

almeno per noi vaccinati. Prima o poi i senatori Questori dovranno esaminare la possibilità, se tutti sono vaccinati, di una diversa regolamentazione (ma è un altro problema). Il Governo aveva Il Governo aveva chiesto una sospensione per esprimere il parere; spero che abbia maturato una decisione.

disegno di legge, che semplifica, come già abbiamo avuto modo di sottolineare nella discussione generale e dopo la relazione del relatore, il procedimento elettorale. Non è sicuramente un disegno di legge che scalda il cuore degli italiani, ma comunque è un provvedimento che semplifica molti aspetti del procedimento elettorale e li allinea alla disponibilità della tecnologia, cosa che fino ad ora non era avvenuto. Inoltre, per quanto riguarda soprattutto il contenuto dell'articolo 4 circa la pubblicazione dei certificati del casellario giudiziale,

quello relativo al deposito del simbolo elettorale, che potrà essere presentato anche in formato digitale e non più solo in formato cartaceo (come avveniva fino ad oggi). Inoltre, le autenticazioni delle firme saranno possibili anche tramite avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato tale disponibilità al proprio ordine;

della pubblicazione dei certificati del casellario giudiziale. Prima tale adempimento era tutto a carico dei partiti, che dovevano richiedere i certificati al tribunale e poi li dovevano pubblicare sul proprio sito.

Se il tribunale non manda il certificato, il partito si ritiene non responsabile di questo mancato invio e fa fede la richiesta fatta al tribunale attraverso la posta certificata. Si tratta, quindi, di una serie di elementi che semplificano il procedimento elettorale, rendono più facile la presentazione delle liste, evitano il sovraffollamento degli uffici e tengono conto dell'importanza delle tecnologie attuali, come la posta elettronica certificata, certificata, per snellire le comunicazioni, evitando gli affollamenti degli uffici, le difficoltà oggettive che spesso determinano ritardi nella presentazione delle liste, i ricorsi e tutto ciò che va a intasare gli uffici pubblici

in Commissione affari costituzionali, approvando convintamente le modifiche intervenute. Queste rendono più omogeneo e più ampio il campo di intervento rispetto al testo iniziale, che riguardava invece soltanto la comunicazione, sempre via PEC, dei rappresentanti di lista. Oltre a quella norma ce ne sono tante altre, come ho detto, che permettono di semplificare il procedimento preelettorale. È per questo motivo che Italia Viva-P.S.I. voterà a favore dell'approvazione di questo disegno di legge. il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore di questo disegno di legge, anche in virtù delle modifiche che sono state introdotte con gli emendamenti che abbiamo appena votato. Ogni procedimento elettorale deve essere improntato al principio di efficienza e semplicità e, soprattutto, al principio della conservazione degli atti che comunque raggiungono lo scopo cui sono destinati. A volte, la prevalenza della forma sulla sostanza porta al formalismo che, come sappiamo, è nemico della democrazia e non suo alleato. La semplicità è la cifra con la quale dobbiamo lavorare per rendere il procedimento elettorale il più chiaro ed efficiente possibile. Certamente, con queste modifiche andiamo in questa direzione, anche se, a nostro parere, si sarebbe potuto fare ancora di più. Purtroppo, però, alcune delle nostre proposte in Commissione sono state ignorate e disattese dalla per cambiare. Eppure il nostro atteggiamento rimane costruttivo e propositivo, nonostante questa maggioranza continui a ritenersi autosufficiente e, a volte, continui a dimostrare

che ancora oggi, nonostante stiamo discutendo di modificare il procedimento elettorale e alcune sue regole, non conosciamo la data precisa del voto amministrativo del prossimo autunno. Sappiamo infatti che si voterà in una finestra che va dal 15 settembre al 15 ottobre, ma non sappiamo ancora la data precisa. Questo è molto grave, signori del Governo e della maggioranza, perché manca poco manca poco tempo e c'è Ferragosto di mezzo. La democrazia ha i suoi tempi: comprimerli in questo modo non è un servizio alla democrazia, tanto più che sono rinviate anche le elezioni provinciali, in attesa dei ballottaggi, che si svolgeranno ancora più avanti. Quindi ci sono istituzioni importanti, che rispondono ai bisogni dei cittadini sul territorio, che sono bloccate e non possono rinnovarsi, a causa di questi tempi

consapevole che, se anche voi non ci ascoltate, gli italiani fortunatamente ci ascoltano sempre di più.

a inserire tra le priorità del nostro impegno legislativo la rimozione di alcune parti, poco ragionevoli, della normativa riguardante il procedimento elettorale e a farlo nel segno della semplificazione e dell'equità, ricercando, attraverso un lavoro importante dei comitati ristretti, punti di intesa tra forze politiche differenti. In questo clima, ci è stato possibile raggiungere risultati significativi - quello di oggi è uno, ma non è il solo - e credo che questo vada sottolineato e debba essere ritenuto un esempio da seguire, anche per portare a casa altri risultati, nell'interesse comune. È evidente che

delle operazioni di deposito dei nomi dei rappresentanti di lista. In generale, si rende più fluido il rapporto tra pubblica amministrazione

dare un'organizzazione più semplice all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, introducendo la possibilità per i partiti

In quale solco si inseriscono dunque questi interventi legislativi, che hanno avuto l'appoggio unanime della nostra Commissione e che, come tali, sono approdati in Aula? Si inseriscono in un contesto che, negli ultimi tempi, impegnati a fare altri aggiustamenti importanti della disciplina elettorale. Cito soltanto quello riguardante le norme che disciplinano la validità delle elezioni

degli iscritti nell'elenco dei residenti all'estero nella platea degli aventi diritto; sapevamo quindi di avere grandi problemi, in molti casi, a garantire la possibilità di elezioni decidenti. Con l'intervento che è stato fatto e che quest'Assemblea ha di recente approvato, abbiamo inserito un elemento di razionalizzazione importante, come lo è stata l'azione contro le liste fantasma. Vorrei dire che con lo stesso spirito speriamo di arrivare presto all'approvazione in Commissione di una legge che ci consentirà, per la prima volta, di recepire in tempi molto rapidi una sentenza monito della Corte costituzionale (la (la n. 48), che, sempre riguardo al procedimento elettorale, ci ha ammonito sull'esistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale per chi presenta candidature alle elezioni per la Camera e per il Senato, che, diversamente da quanto accade per l'elezione di altri organismi rappresentativi, si trovano privi di un giudice al quale poter rivolgere istanze e obiezioni per quello che riguarda le operazioni di carattere prettamente pre-elettorale. Stiamo approfondendo la questione, abbiamo ascoltato molti esperti e contiamo, con lo stesso metodo con cui abbiamo potuto definire il provvedimento in esame, di arrivare a un risultato anche su questo fronte. Devo dire che sono determinanti il confronto tra le forze politiche e l'apporto che in questi comitati ristretti ci ha sempre correttamente fornito il Governo. Considero tutto quello di cui ho parlato finora di buon auspicio anche per riforme più grandi e importanti, che mi auguro la Commissione possa affrontare e che si possono innestare su questo clima di condivisione e di consenso ampio che ha caratterizzato questi provvedimenti e che sarebbe bene riscontrare sempre ogni volta che si parla di regole del gioco. Ribadisco l'orientamento favorevole del Partito Democratico al provvedimento e ringrazio ancora tutti i colleghi della Commissione per il fattivo contributo che hanno fornito al buon esito dei nostri lavori di approfondimento e di costruzione della normativa.

di prendere ogni volta una questione e di operare semplificazioni per settore, forse ci troveremmo davanti a risultati molto più immediati e meno complicati avremmo la possibilità di analizzare meglio nel campo in cui operiamo. Invece, purtroppo, continuiamo ogni anno, perché è diventato di moda, a fare decreti di semplificazione su tutto l'universo mondo; non semplifichiamo la vita dei cittadini. In questo caso, certamente operiamo in un campo ristretto e limitato, che però è importante, ossia quello della partecipazione democratica

di partecipazione dei cittadini, che liberamente si associano e magari liberamente vogliono presentarsi alle elezioni.

di innovazione e rivoluzione digitali e spesso non ci rendiamo conto di avere una serie di norme, soprattutto nella pubblica amministrazione,

di più elementi di certezza dal punto di vista della legalità e della trasparenza, che nel procedimento e soprattutto negli adempimenti pre-elettorali sono un requisito Attraverso gli articoli da 1 a 5 si introducono, quindi, queste misure di semplificazione. In materia di deposito dei contrassegni elettorali, per la verità, siamo tutti un po' romantici

novità che semplificano, aiutano e danno certezza, perché spesso ci sono problemi anche nel deposito dei contrassegni. In questo modo, a mio avviso, semplifichiamo bene.

dei cittadini possa essere non solo semplificata, ma supportata. Non c'è bisogno che tutti abbiano chissà quali risorse, ma i cittadini che vogliono lavorare per costruire un disegno di legge di iniziativa popolare o per

legge stia a testimoniare che è un lavoro che si può fare e in questo caso semplifica la vita certamente delle forze che si presentano alle elezioni, ma incentiva anche molto la partecipazione - perché la semplifica - dei cittadini alle elezioni, alla vita politica e anche all'iniziativa popolare. Non si tratta soltanto di un ammodernamento, di un adeguamento al processo di digitalizzazione, ma è un ulteriore elemento che, nel riaffermare e nel garantire ancor di più i principi di trasparenza e legalità di tutto il procedimento elettorale, aiuta molto e facilita la partecipazione politica. Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole a Signor Presidente, onorevoli rappresentante del Governo e colleghi, desidero fare una premessa alla mia dichiarazione di voto su questo provvedimento e voglio dare atto

è stato instaurato questo criterio, sicuramente per merito del presidente Parrini, che ringraziamo, ma anche per senso di responsabilità di tutti i rappresentanti. Quello in esame è l'ennesimo provvedimento che viene licenziato all'unanimità all'interno del comitato ristretto e quindi della Commissione e che si appresta ad avere il voto unanime di tutta l'Assemblea. Il presidente Parini ha citato il semplificazione della raccolta delle firme del *quorum* di validità per le elezioni e ha anticipato l'adeguamento al monito della Corte costituzionale; citare anche l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, che è stato un lavoro laborioso, ma al cui termine si sono trovate una sinergia e una sintesi che hanno soddisfatto tutti e credo che il Parlamento abbia fatto un ottimo lavoro. Non voglio tornare sulle semplificazioni che questo provvedimento ha portato e che il Senato si appresta a varare, con l'auspicio che anche la Camera dei deputati lo esamini in tempi rapidi, perché possa essere utilizzato già al prossimo turno

Signor Presidente, nella semplificazione delle varie procedure e anche nel solco di una campagna di digitalizzazione che il Governo e questa maggioranza hanno lanciato (che mi auguro sia portata a termine con rapidità,

ai rappresentanti dei partiti di richiedere i certificati elettorali per PEC e obblighiamo i Comuni a rispondere per PEC entro

che c'era una sanzione, ma non una delega al partito. Il provvedimento in esame faculta invece il rappresentante del partito sia nazionale, sia di lista civica a sostituirsi al candidato negligente nella richiesta del certificato penale. E qui c'è l'anomalia, che non si spiega,

quando si arriva agli oneri dei rappresentanti del Ministero della giustizia (nella fattispecie, i dipendenti del casellario giudiziario)

che andrebbe semplificato e di molto, in quanto piuttosto che avere file di persone che vanno quotidianamente a richiedere il certificato penale, con un semplice *click* (rispettando la trasparenza, la legittimazione, la delega e quant'altro) sarebbe stato possibile mandare

Mi auguro che prima o poi si ponga attenzione a questo problema e che ci sia un momento di riflessione, discussione e approfondimento. Le cose non possono andare sempre in questa maniera: il Parlamento non si può fermare di fronte alle ingiustificate

Mi auguro che i nostri rappresentanti all'interno del Governo si facciano portatori di questa situazione e di questo grido di dolore che lancia il Parlamento, dopo aver consumato ore e giorni per trovare sintesi complicate e delicate, ma necessarie, si deve poi fermare di fronte a un ingiustificato rifiuto. Infatti, non vi è una giustificazione valida per cui il casellario giudiziale non possa rispondere per PEC, così come fanno tutti gli altri uffici e gli stessi cittadini che chiedono certificati e svolgono attività.

soprattutto oggi, quando si annunciano decine di migliaia di assunzioni che devono servire proprio per digitalizzare il nostro sistema e renderlo più veloce e rispondente alle esigenze dei tempi moderni. Esprimiamo quindi un voto favorevole ringraziando il collega Lanzi che ha lanciato la pietra nello stagno e ha dato immediatamente disponibilità, quando gli ho chiesto di inserire norme aggiuntive, sempre nel solco della semplificazione. Pur di ottenere un risultato,

è il secondo in pochissimo tempo che è stato trattato e concluso dalla 1a Commissione con esito molto favorevole, non solo per il risultato concreto e formale, ma anche per la modalità di lavoro. Mi riferisco a quelle del comitato ristretto, cui ha partecipato il collega Augussori, che già durante la discussione generale ha spiegato nei dettagli gli articoli del provvedimento.

semplificazioni, che vanno a migliorare davvero il funzionamento della macchina pubblica e a facilitare il lavoro dei cittadini, che in questo caso si trovano nelle vesti di potenziali candidati o di persone che all'interno dei partiti gestiscono le operazioni pre-elettorali o anche incaricati dell'amministrazione pubblica che riescono a velocizzare il proprio lavoro grazie a queste norme

dire. Se riusciamo a portarci a casa un disegno di legge in meno di un mese significa che, quando si parla poco e si lavora tanto, bene in modo collaborativo e cordiale, i risultati ci sono.

così come stiamo facendo noi, da altri colleghi in altre Commissioni per capire quali sono i modi migliori per esercitare il nostro potere

che creavano ansie terribili, soprattutto, come dicevano anche i colleghi, per le liste civiche o per quelle piccole (magari non parliamo dei grandi partiti), perché ci si ritrovava all'improvviso a confrontarsi con la macchina della burocrazia, con cui non si aveva mai avuto a che fare

dare la comunicazione al sindaco per poter fare l'autentica delle firme; semplicemente è in suo potere autenticare le firme come consigliere comunale. Si realizza poi una semplificazione nella richiesta dei certificati elettorali: è possibile farne sia

nonostante a volte si riescano a ottenere bei risultati, anche grazie alla collaborazione tra di noi, si prova sempre un po' di amarezza, quando ci si scontra con problemi interni relativi proprio al funzionamento burocratico dei vari Ministeri, uffici e funzionari.

insormontabile per il progresso di questo Paese, dovremmo innanzitutto cercare di fare in modo che non lo sia neanche per il lavoro di questo Parlamento.

oggi, con l'approvazione di questo disegno di legge a mia prima firma, arricchito dal valido contributo di più colleghi, tagliamo un importante traguardo, portando a compimento un percorso durato solo poche settimane, grazie all'intesa tra tutti i Gruppi. Si tratta di uno dei pochi disegni di legge di iniziativa parlamentare approvati e questo la dice lunga su come si debba migliorare, invertendo la tendenza. Il Parlamento torna a svolgere il ruolo affidatogli dalla Costituzione, occupandosi e modificando di propria iniziativa alcune anacronistiche disposizioni del nostro ordinamento. La semplificazione e la digitalizzazione previste da questo testo riguardano tutte le procedure preelettorali, ma ancor più importante è il fatto che l'approvazione di questo disegno di legge segni l'adozione - oserei dire Adesso i partiti non avranno più scuse. Infatti, tra le tante migliorie, le forze politiche potranno richiedere il certificato penale prima di candidare gli aspiranti: modello 5 Stelle! Noi da sempre facciamo così; non è mai troppo tardi per seguirci in questi percorsi e vi diamo il benvenuto. Come ho già espresso in sede di discussione generale, l'approvazione di questo disegno di legge non può considerarsi un risultato scontato, perché esso semplifica, senza colore politico, un tema non eticamente impegnativo, come invece lo sono, senz'altro, l'eutanasia e la cannabis terapeutica, di cui quest'Assemblea dovrebbe presto occuparsi. un disegno di legge semplice, ma ciononostante, senza la mia insistenza, l'impegno del relatore, senatore Vincenzo Garruti, il sostegno di tutti, a partire dal presidente della 1a Commissione, senatore Dario Parrini, del senatore Luigi Vitali della capogruppo, senatrice Maria Laura Mantovani, e i consigli del presidente, senatore Roberto Calderoli, saremmo ancora lontani dalla sua approvazione. Infatti, se dal lato politico abbiamo trovato ampie sponde da parte anche dei nostri Sottosegretari, *in primis* Carlo Sibilia, che ha seguito il provvedimento, non posso che rilevare il solito ostracismo burocratico da parte di talune strutture ministeriali, che molto spesso tentano di rallentare le forti istanze di cambiamento provenienti dalla società civile, anche per il tramite della politica. allora rimarcare la tanto declamata separazione tra politica e amministrazione, oggetto di numerosi interventi legislativi, ma ancora oggi non del tutto attuata. È inaccettabile quest'ostracismo. Considerando che le dichiarazioni di voto hanno valenza di atto preparatorio, è stato presentato un emendamento, appena approvato, per introdurre il termine di cinque giorni per consentire al tribunale di trasmettere i certificati al richiedente, con l'auspicio che i tribunali utilizzino per la consegna dei certificati tutti i canali telematici a loro disposizione, a partire dalla PEC, recependo il parere della Commissione referente. Tornando però alle semplificazioni in discussione, è chiaro che sulla medesima materia si può fare ancora di più. Mi riferisco ad altre proposte già depositate, che avremo l'occasione di tradurre presto in norme concrete, Senato 862, un disegno di legge a prima firma della senatrice Felicia Gaudiano, elaborato per scongiurare comportamenti fraudolenti posti in essere da rappresentanti di lista, volti ad esprimere più volte il proprio voto nell'ambito della medesima consultazione elettorale. Mi riferisco anche all'emendamento 5.1, presentato dal senatore Sergio Vaccaro, che, se approvato, avrebbe introdotto ulteriori semplificazioni nel procedimento di nomina degli scrutatori. presidente Parini, come ha detto poco fa, raccolga la sfida e chiudiamo insieme anche su queste osservazioni, senza indugio. In conclusione, mi auguro adesso che anche la Camera dei deputati mostri la stessa sensibilità sul tema e proceda in tempi altrettanto brevi alla definitiva approvazione di questo disegno di legge. Esso dev'essere operativo per le elezioni amministrative suppletive del prossimo autunno, altrimenti tutto il nostro impegno verrebbe vanificato. Concludendo, felici per il lavoro svolto da questo ramo del Parlamento, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

Signor Presidente, colleghi, non deve sorprendere l'istituzione di una Commissione di inchiesta nella materia del gioco. Anzi, testimonia la grande attenzione della politica rispetto ad un settore caratterizzato da molti aspetti, che giustificano punti di vista differenziati, se non addirittura antitetici. Il mestiere della politica è proprio questo: ascoltare, verificare le diverse posizioni e poi tentare di fare una sintesi. Questo schema operativo è già stato messo in campo dalla Commissione finanze nell'esaminare il documento presentato dai senatori del Gruppo Italia Viva, a prima firma del collega senatore Marino. La Commissione ha condiviso da subito l'iniziativa, concentrando la fase emendativa sulle disposizioni che potevano indurre in un errore di prospettiva. L'oggetto dell'inchiesta non è il gioco pubblico in Italia, ma il gioco illegale e le eventuali disfunzioni del gioco pubblico. Infatti, è opinione prevalente e condivisa, anche tra i Gruppi parlamentari più critici e sensibili alle conseguenze sociali della diffusione del gioco d'azzardo, che il comparto del gioco è una componente economica e produttiva importante, con profili occupazionali e di gettito erariale meritevoli di grande attenzione e certamente non può essere oggetto *tout court* di un'inchiesta parlamentare o amministrativa, anche in relazione all'esecuzione delle concessioni, anche verificando l'eventuale verificarsi di sovrapposizioni e antinomie nell'azione di contrasto al gioco illegale. Particolare attenzione sarà posta nell'evitare che i compiti dell'istituenda Commissione possano sovrapporsi a quelli di altri organismi di inchiesta, in particolare con la Commissione antimafia, il cui lavoro di approfondimento è precipuamente

dal primo all'ultimo, perché da ciascuno è venuta una grande disponibilità al dialogo, all'ascolto e alla collaborazione, e questo disegno di legge è il frutto di questo clima collaborativo.

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signori rappresentanti del Governo, con questo provvedimento riprendiamo idealmente un percorso interrotto nella scorsa legislatura; un percorso irto di ostacoli quale si sovrapponevano sensibilità diverse: c'è chi optava per una riforma sistemica e chi invece preferiva l'analisi settoriale. In tal modo si sovrapponevano

i due profili prioritari erano quelli che afferivano alla Commissione finanze e al tema della Commissione sanità. In realtà, il percorso era molto più lungo partiva dalla legge di delega fiscale, la legge n. 23 del 2014, dove, all'articolo 14, si davano indirizzi perché vi fosse una raccolta sistematica della disciplina in un codice di disposizione dei giochi. Si ipotizzava poi il riordino del prelievo erariale, interventi volti a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi, nonché interventi volti a recuperare dal disturbo del gioco d'azzardo, il DGA, quello che noi volgarizziamo in ludopatia, le persone maggiormente esposte. Cito solo questi, perché sono alcuni dei temi più significativi. Purtroppo questa norma fu uno dei cinque punti inattuati della delega fiscale, insieme a quello del catasto, della giustizia tributaria, della fiscalità ambientale e della riscossione degli enti locali. La delega scadeva il 27 giugno 2015. Preso atto del fallimento dell'attuazione della delega in materia, la legge di stabilità del 2016 interveniva, all'articolo 1, dando disposizioni che, in sede di conferenza unificata Stato-Regioni, venissero definite: le caratteristiche dei punti di vendita dove si raccoglie il gioco pubblico; criteri di distribuzione e di concentrazione territoriale dei punti di vendita, ma anche la tutela della salute, la tutela dell'ordine pubblico, la tutela della pubblica fede dei giocatori e, naturalmente, la tutela dei minori di età. Il 5 maggio 2016 iniziò un confronto sulla regolazione dei giochi, con gli enti locali e con la Commissione antimafia: sensibilità particolari, anche rispetto alle mozioni approvate dal Parlamento e ai disegni di legge parlamentari. In altre parole, lo Stato voleva ragionare sulla distribuzione dell'offerta e regolarla, perché l'aumento dell'offerta, che era la risposta che veniva data al gioco illegale, trovava una reazione, da parte degli enti locali, che ravvisava un effetto di emergenza sociale. Su tutto, chiaramente, dominava la mancanza di un quadro regolatorio nazionale, a fronte del fatto che nel 2016 il gettito per l'erario fosse di ben 10,5 miliardi di euro. Contemporaneamente, a fronte di quanto veniva vissuto come un procedere claudicante da parte dell'Esecutivo di allora, vennero presentati diversi disegni di legge, che, fondamentalmente, solo al Senato si aprirono in due filoni: uno faceva riferimento al disegno di legge presentato dal senatore Mirabelli, che chiedeva anche la procedura d'urgenza *ex* articolo 77 del regolamento del Senato e che aveva un carattere ampio, trattandosi di disposizioni in materia di riordino dei giochi. Ve ne erano altri. Per citarne solo alcuni, quello del senatore Endrizzi, che è presente in Aula, ma anche quelli della senatrice Albano e del senatore Crosio, che invece ragionavano più sulla pubblicità dei giochi. Si apriva addirittura un conflitto di attribuzioni tra Camera e Senato, che veniva risolto dai due Presidenti delle Camere ponendo la trattazione della materia in capo al Senato. Quando sembrava che, finalmente, l'*iter* parlamentare fosse sulla rampa di lancio,

la Conferenza unificata, sarebbe saggio sfruttare l'occasione migliore. Dopo un dibattito parlamentare su questo tema, il Parlamento decise di fare un passo indietro e di lasciare mano libera al Governo, il quale firmava l'intesa in Conferenza unificata il 7 settembre 2017. Intesa che, però, non veniva rispettata proprio da parte di alcuni sottoscrittori.

Quindi, se si uniscono la narrazione storica di quanto è successo, l'incremento verticale del fenomeno del gioco in generale e la dimensione crescente del gioco illegale, che ha subito un picco proprio in occasione della pandemia e che ha costretto alla diminuzione dell'offerta del gioco legale, a fronte delle necessarie chiusure, si capisce il perché dell'opportunità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico.

delle fonti, capire quale sia il ruolo svolto effettivamente dall'eventuale presenza di soggetti criminali in relazione al riciclaggio di denaro, alla manipolazione dei terminali di gioco, ma anche alla creazione di una rete parallela dell'usura in cui finiscono molti dei soggetti deboli che vengono risucchiati da questo vortice, verificare quale sia l'impatto delle trasformazioni tecnologiche del sistema, a partire dal gioco *on-line*, che ha finito per assumere un ruolo preponderante in alcuni settori, nei quali si dovrà intervenire sotto il profilo normativo, normativo, e verificare l'efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli e al contrasto della diffusione del disturbo da gioco d'azzardo. Colleghi, non elenco i contenuti, che vedrete dettagliati nell'articolo 3 del testo al nostro

Questo è il quadro: adesso è importante che questo lavoro di analisi venga fatto senza il velo del pre-giudizio, nel senso etimologico del termine e con un atteggiamento che, permettendomi di prendere a prestito le parole di Tacito all'inizio degli "Annales", sia veramente *sine ira et studio,* ovvero senza animosità e simpatia.

Con questo spirito costruttivo, il Gruppo Italia Viva dice un convinto sì all'approvazione della proposta di inchiesta parlamentare

Non possiamo però non ricordare all'Assemblea, ai colleghi della maggioranza, ai colleghi del centrodestra, agli amici della Lega e di Forza Italia, se c'era bisogno di questa Commissione, riteniamo da tempo ci sia bisogno anche di una Commissione sul tema del Covid-19 e della pandemia,

arrivare anche per un tema che molti italiani da tempo attendono venga affrontato, con identica serietà e impegno. Detto questo, vorrei fare delle considerazioni anche terminologiche, a proposito della Commissione che dal titolo vediamo essere una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto al gioco illegale. Bene, a livello terminologico credo sarebbe stato più corretto - lo dico anche per far capire

e di una Commissione di indagine su quello che è invece il fenomeno fisiologico, cioè sul gioco pubblico e legale. Con questo spirito ci approcceremo a questa Commissione, che sicuramente dovrà essere d'inchiesta sul fenomeno in crescita - ahimè - del gioco illecito e che dovrà essere invece, in modo costruttivo, di indagine sul gioco pubblico e legale. legale. Una distinzione terminologica che non è formale, ma assolutamente sostanziale.

la problematica delle ludopatie, che certamente è presente in tutti noi, la problematica dell'illegalità e delle mafie, sulle quali tornerò, e le problematiche - permettetemelo di dire anche con un po' di *pathos* - del gioco pubblico. Tali problematiche hanno riguardato un settore composto da decine di migliaia di piccole imprese e da oltre 150.000 occupati, che stanno soffrendo tredici mesi di *lockdown*. Non dimentichiamoci che i sacrifici che sono stati spesso erroneamente imposti, come abbiamo più volte sottolineato, a tante imprese italiane, ai bar, ai ristoranti e alle palestre, sono sacrifici che vedono negli operatori del gioco pubblico, cioè nei concessionari dello Stato (non dimentichiamocelo), coloro che più sono stati colpiti e meno sono stati aiutati. Quindi ricordiamoci - anche la Commissione se lo dovrà ricordare - di decine di migliaia di operatori del gioco pubblico e di oltre 150.000 occupati nel settore. Venendo quindi ai singoli aspetti, c'è il tema della ludopatia. Quando si approccia il fenomeno del gioco,

Questo è il primo aspetto che dobbiamo prendere come riferimento quando affrontiamo il tema delle ludopatie. A questo riguardo, dobbiamo subito dire che la patologia, cioè il degenerare della passione per il gioco, trova una barriera prima di tutto negli operatori del gioco pubblico, perché questi sono gli unici che devono attenersi alle regole date, che possono controllare che i minori non giochino e che possono controllare i fenomeni degenerativi. In sostanza, le normative, le limitazioni e le tutele che vogliamo porre e che abbiamo posto per salvaguardare le persone vedono negli operatori legali i primi artefici e sostenitori. Viceversa, laddove, spesso anche in modo insensato, le le Regioni hanno provocato di fatto le chiusure degli operatori del gioco legale (penso ad esempio al Piemonte o all'Emilia-Romagna),

che prosperano sulla chiusura del gioco legale, che non si attendono altro che norme restrittive e proibizionismo crescente, perché lì guadagnano e brindano. Questo dobbiamo dircelo chiaramente.

Sarà una strada - che ritengo non auspicabile - di ghettizzazione del gioco, magari nelle grandi sale, dove naturalmente il giocatore viziato, patologico e che si isola trova

Questi sono temi sui quali dovremo ragionare, anche nell'ottica di una riforma e quindi della tutela dei nostri concittadini, che devono approcciarsi a questo mondo in modo naturale e non perverso.

quindi l'illegalità da combattere attraverso una riforma del gioco pubblico: per questo prima parlavo di indagine sul gioco pubblico. Arriviamo dunque in modo costruttivo a una riforma che sia nell'interesse vero del Paese e nel contrasto alle mafie e all'illegalità, che invece, ribadisco, con le censure *tout court*, trovano solamente conforto. Questi sono dati pubblici, riscontrati peraltro dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza.

e, dall'altra, se garantire il monopolio delle multinazionali, perlopiù straniere, oppure dare lavoro alle piccole imprese italiane. Questa è un'altra discriminante che per Fratelli d'Italia è importante e su cui chiederemo a tutti ausilio. Ribadisco e chiudo, signor Presidente, chiederemo a tutti ausilio sulla tutela dei nostri concittadini, sulla lotta a ogni forma di

molto importante per l'economia del Paese, un settore che ha bisogno davvero di

Troppe cose si sono susseguite. Manca una riforma organica del settore stiamo parlando di un settore importante, che garantisce otto miliardi all'anno di entrate allo Stato italiano, ma che è anche fortemente permeabile alla criminalità e alla illegalità. Molte sono le inchieste che abbiamo visto susseguirsi da Nord a Sud in questi mesi e in questi anni, che hanno visto la criminalità organizzata penetrare il gioco legale o gestire il gioco illegale. Rispondere a tutto questo significa valorizzare, come è giusto fare, l'importanza del gioco legale, mantenere un gioco legale anche per contrastare l'illegalità, ma bisogna sapere che ciò non Bisogna verificare i capitali delle società legali: chi investe nel gioco legale? creare regole più ferree e più forti rispetto al gioco *online*, che oggi è un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più. Bisogna stabilire regole ferree come quelle che hanno garantito, il provvedimento che abbiamo approvato nella scorsa legislatura, la possibilità, come era necessario, di collegare tutte le *slot machine* e tutti gli apparecchi VLT da remoto, per impedire quelle truffe ai consumatori che venivano perpetrate modificando le schede

Immagino che siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna contrastare le ludopatie e sappiamo che il gioco, anche quello legale, produce in alcuni soggetti dipendenza. Sappiamo bene che ci sono famiglie che sono state rovinate dal gioco, e non da quello illegale. Bisogna contrastare le ludopatie, bisogna stabilire regole ferree nel funzionamento, ad esempio, delle VLT e delle *slot machine*, per evitare che le persone si rovinino. lenti di gioco, la possibilità di giocare somme di denaro inferiori a quelle che si possono giocare. Se vogliamo contrastare le ludopatie, dobbiamo ridurre domanda e offerta di gioco.

necessaria la tessera sanitaria per poter giocare nelle sale giochi, con l'obiettivo di garantire anche una verifica, di aiutare le persone più predisposte

Dopodiché questo non si può fare se, mentre da una parte riduciamo domanda e offerta di gioco, dall'altra mettiamo nel bilancio dello Stato più soldi

che non possiamo neanche pensare di tutelare un settore economico importante come quello delle aziende che offrono

trovate a fronteggiare una situazione di incertezza costante, di cambio continuo delle regole e di impossibilità di prevedere il loro futuro e - aggiungo - anche di trovare uno Stato che le aiuti nel momento in cui cui si chiede loro di riconvertirsi e fare altro proprio per ridurre domanda e offerta di gioco. Penso che per queste ragioni serva una riforma di riordino complessivo del settore e mi auguro che il Sottosegretario che ha la delega

pochi giorni prima della nuova legislatura, quando, dopo un lungo lavoro, si era finalmente trovata una quadra. Chiederei al Sottosegretario di ripartire da lì,

La Commissione può essere utile per fungere da sprone, dare argomenti e costruire approfondimenti, ma noi abbiamo bisogno di una legge di riordino.

in merito all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto al gioco illegale. In Italia il gioco d'azzardo coinvolge circa 10 milioni di persone: dalle scommesse *online* fino alle *slot machine*. I malati di ludopatia sono 1,3 milioni, come acclarato dall'osservatorio nazionale sul contrasto La ludopatia è una piaga sociale anche peggiore dell'alcolismo e della tossicodipendenza. Come ho già avuto occasione di affermare in Commissione finanze oltre alle lotterie istantanee vengono istituite anche commissioni di inchiesta lampo istantanee e ne sono lieto. Mi permetto però di ricordare - lo dico senza acrimonia - che il 22 maggio 2018 (quindi oltre tre anni fa) avevo presentato la proposta di legge n. 411, la terza a mia prima firma dopo le norme a tutela e garanzia del diritto di proprietà della prima casa quest'ultima, purtroppo proprio oggi la Consulta ha dichiarato incostituzionale la seconda proroga, dal primo gennaio al 30 giugno 2021, della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa, oltre alle disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni che comportino il vincolo di obbedienza, come richiesto da logge massoniche o da associazioni fondate sul giuramento o sul vincolo di appartenenza. La proposta di legge n. 364, norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, assegnata il 20 ottobre 2018 alle Commissioni finanze e sanità, nonostante i solleciti, giace impolverata nei cassetti delle Commissioni. Certo, la pandemia ha cambiato le cose. Secondo l'Istituto superiore di sanità (ISS) la presa di coscienza di essere ludopatici con il *lockdown* è aumentata; stando a casa sono in crisi di astinenza. L'impossibilità di giocare d'azzardo per una persona con un disturbo specifico può causare un aumento del livello di stress, inquietudine, aggressività disturbi del sonno, al punto tale da inasprire le relazioni sociali di convivenza. Dunque, improvvisamente, in tanti si sono accorti di avere una dipendenza. La situazione è gravissima soprattutto quando i ludopatici giocano. Le persone affette da ludopatia solitamente stabiliscono con il gioco un rapporto esclusivo e altamente coinvolgente. L'elevato livello di eccitazione li spinge a trascurare famiglia, affetti e lavoro, per non parlare dei soldi sottratti alla quotidianità della famiglia. In base al Libro Blu, redatto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in Italia ogni anno le giocate superano i 110 miliardi di euro, una cifra equivalente a due gigantesche manovre finanziarie. È come se ogni italiano scommettesse un totale di 1.780 euro l'anno

per quanto riguarda il gioco fisico, del 16 per cento invece se ci si riferisce al gioco *online*. I cosiddetti *poker cash* fanno la parte del leone e si tratta di giochi in cui c'è sempre un unico vincitore: la società che promuove il gioco. Il giocatore perde sempre, a volte arriva a ridursi sul lastrico; ma c'è di più: il gioco d'azzardo non riduce soltanto il tenore di vita del ludopatico e del suo nucleo familiare; a rimetterci è anche l'economia reale a cui vengono sottratte risorse preziose. Il giocatore compulsivo limita infatti le proprio capacità di spesa con evidenti danni al circuito economico e commerciale e, in più, colpisce soprattutto le fasce più basse della popolazione, le persone con minor grado d'istruzione, quelle con i lavori precari.

Inoltre sono in allarmante aumento le applicazioni per telefoni cellulari e *tablet* che offrono centinaia di giochi d'azzardo, scaricabili gratuitamente anche nella versione per bambini con immagini e *format* accattivanti. Sempre più minorenni utilizzano quotidianamente telefoni cellulari e *tablet* da cui possono accedere alle applicazioni del gioco d'azzardo. Tra i giovanissimi è altissimo il rischio di sviluppare dipendenza dal gioco d'azzardo. È proprio lo Stato il primo responsabile di questo disastro sociale. Gli apparecchi di intrattenimento, ovvero *slot machine* e *videolottery* si confermano i più utilizzati con il 63 per cento delle giocate complessive su rete fisica. Seguono le lotterie, comprese quelle istantanee, i cosiddetti «gratta e vinci», con il 12,4 per cento, e le varie tipologie di Lotto, con il 10,8 Va bene quindi, colleghi, signora Presidente, indagare sul settore del gioco pubblico e sul contrasto al gioco illegale, ma la ludopatia ed i costi sanitari e sociali il gioco che si accanisce sui più deboli con la complicità dello Stato avrebbe meritato maggiore attenzione. Il gioco d'azzardo, che per Camillo Benso di Cavour era la tassa volontaria sugli stolti, la tassa sugli imbecilli, si accanisce sui più deboli, proprio coloro che lo Stato, tramite la Costituzione, dovrebbe proteggere, quindi non dovrebbe Bisognerebbe cambiare paradigma, iniziando a trattare il gioco d'azzardo con lo stesso approccio con cui si affronta la droga, senza nascondere la testa sotto la sabbia facendo finta, per salvaguardare le entrate erariali, di non conoscere i costi sanitari, sociali ed umani che lo Stato biscazziere è costretto a pagare

per chi ha vissuto l'avventura di una riflessione intensa, accesa, prolungata nel tempo, capace di sollevare problemi di ogni tipo e ordine in merito al gioco d'azzardo, la Commissione di inchiesta arriva un poco come un fulmine a ciel sereno. Tutti noi avremmo voluto una legge quadro sul gioco d'azzardo; tutti noi avremmo voluto poter discutere su una legge nella sua struttura organica. Oggi, invece, con la Commissione d'inchiesta ci troviamo a intervenire in maniera chirurgica o comunque comunque più simile al lavoro che fa un medico quando interviene su un corpo che considera già malato, infettato. Istituire una Commissione d'inchiesta, infatti, significa assumere già in premessa che ciò che c'è non va bene; significa assumere in premessa una visione in cui gli elementi gli elementi di pericolosità di quello che in questo momento stiamo facendo sono insiti nella struttura stessa, quella che possiamo considerare l'infrastruttura del gioco d'azzardo.

attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, che a sua volta lo esercita attraverso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che a sua volta lo esercita attraverso i suoi concessionari, che a loro volta lo esercitano attraverso i gestori.

entrate che superano i 14 miliardi; qualche anno fa erano quasi pari a una manovra finanziaria. Oggi non sappiamo più che cosa sarà una manovra finanziaria, quali saranno le sue dimensioni, probabilmente stratosferiche, ma c'è stato un periodo di tempo in cui dal gioco d'azzardo lo Stato ricavava energie importanti per la fiscalità generale e questo creava quel conflitto d'interessi

tutt'al più potrebbe avere un certo interesse a regolamentarlo, ma sempre senza ridurre il gettito fiscale di cui si avvale.

giovedì e venerdì, quando al Ministero della salute si cercherà di fare il punto sulla salute mentale. Vedremo allora quanto sono scarsi gli investimenti che si fanno, sotto tanti aspetti, anche per controllare il fenomeno drammatico delle dipendenze. La ludopatia è una dipendenza del tutto particolare, perché è senza materia: la dipendenza dall'alcool ha una materia, che è l'alcool (mi astengo dall'alcool); la dipendenza dal tabacco ha una materia, il tabacco da fumo (mi astengo dal fumo); della dipendenza dalle droghe non ne parliamo nemmeno. Poco fa qualcuno dei colleghi ha invocato il fatto che in quest'Aula noi dovremmo parlare di liberalizzazione delle droghe, cioè di questa spaventosa dimensione che crea dipendenze di tutti i tipi, generi e specie, che a sua volta diventa una fonte di rischio altissimo. rischio altissimo. Cosa fa lo Stato per affrontare la patologia? In che misura si fa carico, per esempio, dei lunghi processi di psicoterapia di cui ci sarebbe bisogno per spostare spostare il centro dell'attenzione di queste persone dal gioco ad altri obiettivi, che riguardano l'affermazione di sé, la propria identità, l'autostima? Fa pochissimo o nulla. Non fa molto di più per nessun altro aspetto della salute mentale, ma su questo fronte preciso non fa nulla. Sapete dove si curano le persone affette da azzardopatia?

a contrarre dipendenza da qualunque oggetto che in quel momento sembri soddisfare la logica del desiderio. Cosa fa lo Stato, che tanto incassa, per rimediare a questi rischi? E non ci sono solo i rischi della salute fisica e della salute mentale; ci sono anche tutti i rischi collegati a quell'impoverimento che è stato denunciato, descritto, quantificato da altri colleghi. Il giocatore, per definizione, è destinato a un processo di impoverimento. Abbiamo romanzi straordinari e bellissimi (non voglio citare ora quello di Dostoevskij, ma ce ne sono anche di più recenti) che descrivono questo demone, che di fatto comporta necessariamente l'impoverimento, non solo materiale - perché queste persone si giocano tutto

una piccola risorsa economica per far fronte a un debito che poi ti salverà, perché tradurrai quella risorsa economica nella tentazione di giocare.

Questa è volontà perversa di creare un danno senza una riparazione; il resto ruota sicuramente intorno alle dinamiche economiche che si cerca di salvaguardare in tutti i modi: qualunque vantaggio, ma senza riduzione del gettito.

fanno un po' sorridere (i 25 milioni per quest'anno e i 70 milioni per gli anni successivi). Mi auguro che, al di là di quelle che possono sembrare chiacchiere, di fatto si abbia il coraggio di affrontare questa che possiamo considerare una moderna piaga della nostra società.

oggi l'Assemblea è chiamata ad approvare la costituzione di questa nuova Commissione parlamentare d'inchiesta. A nostro modo di vedere il lavoro fin qui svolto presenta molteplici aspetti positivi che ci auguriamo andranno ad incidere e a combattere efficacemente alcune odiose problematiche che affliggono la nostra società, da non ignorare o sottovalutare, ma delle quali ci dobbiamo fare carico. Lo scopo principale di questa Commissione è senza alcun dubbio la lotta decisa al gioco illegale. Questo fenomeno è molto complesso e si manifesta in molteplici forme: come ben sappiamo, produce effetti disastrosi per la nostra società; favorisce la criminalità organizzata; crea dipendenza e contribuisce ad aumentare i casi di ludopatia, solo per citarne alcuni. In queste situazioni il ruolo dello Stato deve essere chiaro e non equivoco: oltre ad una ferma condanna del gioco illegale, lo Stato non deve lucrare sulle debolezze dei propri cittadini. I soggetti più deboli, più fragili e più giovani, potenzialmente più a rischio, devono essere tutelati. Si devono mettere in atto tutte le misure che vadano nella direzione di prevenire di evitare un insensato e innaturale aumento della spesa di singoli e famiglie nel gioco, che possa portare ad un impoverimento, o peggio ancora anche a fenomeni di usura. Ci rendiamo conto che il compito non è assolutamente facile: servono equilibrio e buon senso, serve trovare un equilibrio tra la tutela occupazionale, la tutela delle attività che lecitamente operano in questi settori e quella della salute pubblica. Lo Stato deve farsi carico di garantire correttezza nell'offerta e una leale concorrenza tra gli operatori autorizzati. Ci rendiamo conto della diversificazione delle varie attività e della complessità della normazione di ciascuna. Il settore, infatti, è assai vasto: si pensi, a titolo esemplificativo, alla produzione, alla commercializzazione e alla gestione degli apparecchi di intrattenimento, ma anche alla gestione del settore delle scommesse e a quello delle lotterie istantanee. Non è semplice, ma lo Stato deve farsi carico anche dei più deboli. In questo quadro assume importanza prioritaria e va assolutamente sostenuto il ruolo dell'azione pubblica di prevenzione, di cura e sostegno per i soggetti a rischio o affetti da ludopatia, svolta in particolare dagli enti territoriali e dai servizi sanitari. Una Commissione di inchiesta che faccia piena luce su tali problematiche in tutte le loro sfaccettature e possa individuare misure per contrastare il gioco illegale alla radice è un obiettivo che oggi quest'Assemblea raggiungerà anche grazie al nostro convinto sostegno. La Commissione dovrà inoltre farsi carico di dare maggiore ordine e di armonizzare il sistema del gioco legale in Italia, di analizzare e trovare le migliori soluzioni per tutelare interessi legittimi contrapposti al fine di salvaguardare attività legali ed evitare problemi sociali per i più deboli. Riteniamo che il testo oggetto

il gioco pubblico nella dimensione del gioco d'azzardo è stato oggetto negli anni di interventi normativi e di attenzione da parte della società civile. Ne è derivato un dibattito complesso per la diversità di interessi e di attori coinvolti, che specialmente negli ultimi vent'anni ha comportato tesi contrapposte. Sembrano incompatibili le finalità di un comparto che, a fronte di una dimensione economica rilevante, degenera in ludopatia e disagio sociale con una incidenza percentuale che non è accettabile in uno Stato che deve mettere al centro il benessere e la felicità dei suoi cittadini -, in dipendenze e in illegalità diffusa che attrae le mafie e sfugge al controllo di un impatto di regole non sufficienti e - cosa più grave - non adeguate. L'11 settembre 2020, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha presentato i dati ufficiali sul gioco d'azzardo con la pubblicazione annuale che riporta i dati principali: raccolta, spesa, vincite, incassi erariali. L'Italia è il Paese d'Europa in cui si spende di più per il gioco d'azzardo. La raccolta è passata dai 47,5 miliardi del 2008 ai 110,5 del 2019, con entrate statali quest'anno pari a 11,4 miliardi. Degli oltre 110 miliardi di euro puntati nel 2019, più di 46 miliardi di euro arrivano dalle *slot machine,* e poi i giochi derivati dal lotto, i «gratta e vinci», le sale scommesse e il bingo: tutto basato su un'idea di fortuna discutibile, che solo nel caso dei giochi legati allo sport ha un qualche margine di determinazione nella scelta delle variabili da parte del giocatore. Un panorama in cui si muovono migliaia di persone con numeri che crescono ogni anno anche per la quota del gioco *online*. Anche a causa del Covid-19, e quindi delle chiusure delle sale da gioco e delle limitazioni alla circolazione, abbiamo assistito nell'ultimo anno a un fenomeno in atto da tempo, ossia il deciso aumento del gioco *online* rispetto a quello fisico. Addirittura il gioco *online* avrebbe superato il gioco fisico, secondo una recente dichiarazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Questa però per lo Stato non è una buona notizia, essendo il gioco *online* molto meno tassato rispetto a quello fisico. In tempi normali lo Stato incamera 11 miliardi di euro dai giochi fisici e 350 milioni da quelli telematici. Nel periodo del *lockdown* il gioco d'azzardo *online* è ancora aumentato perché non soggetto alle restrizioni, come invece è toccato a quello fisico, e così a fine 2020 il bilancio dell' *online* è di circa 44 miliardi al lordo. Persone di cui non conosciamo i volti: alcuni di essi piano piano si annientano fino a diventare invisibili e fragili quando, perdendo il senso del tempo e del denaro stesso, diventano prede e poi vittime di azioni criminali come l'usura. Il cosiddetto Libro Blu dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha confermato nel 2019 il *trend* di crescita, sconvolto in seguito alle conseguenze della pandemia, che in realtà ha richiamato le riflessioni sul volto disumano di questo settore. Perché più che parti di una teoria economica, le analisi e gli studi sul gioco sembrano un trattato sulla speculazione. I dati Istat sulla povertà italiana, pubblicati qualche giorno fa, ci restituiscono la fotografia di un Paese in grande difficoltà, con 5,6 milioni di persone (circa una su 10) in condizioni di povertà assoluta, cioè con difficoltà ad arrivare alla fine del mese, nonostante misure importanti adottate dagli ultimi Governi, come il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, il reddito d'emergenza, cui aggiungiamo i tanti cassaintegrati, su cui pende l'incertezza del futuro. Non è certo di giustizia sociale che si parla quando si parla di puntate e scommesse. La giustizia sociale agisce contro ogni forma di discriminazione e tutela i diritti imprescindibili di ciascuna persona. Oggi è il valore della persona, della sua fragilità e dei suoi diritti, ad essere minacciato dalla diffusa tendenza a ricorrere esclusivamente ai criteri dell'utilità e dell'avere imposti dall'economia liberista. Forme di Stato e di Governo che attuano politiche sociali fondate su principi transgenerazionali, misurate e misurabili sull'impatto nella vita di ciascuna persona, sono temi ormai diventati protagonisti del cambiamento in atto verso la sostenibilità e lo sviluppo umano integrale. Oggi, in tempi di pandemia, dobbiamo parlare di uno Stato che premia le imprese che creano valore e avviarci verso un modello economico sostenibile, che genera ricchezza e benessere. L'economia dell'azzardo, invece, è costruita su una mega macchina sociale, che estrae valore e non genera ricchezza. Il gioco d'azzardo è un'operazione finanziaria in sé, non dispone di progetto industriale e di economia reale sottostante. Chiediamoci, allora, quali sono i costi reali da computare per rimanere nei temi dell'etica. Ben venga una Commissione di inchiesta che mostri intransigenza sugli affari della criminalità e che abbia una forza generatrice di idee innovative per le politiche sociali correlate. Riflettere sul gioco, dunque, come strumento, riconoscendone le ricadute negative nell'utilizzo illegale e non controllato. Non siamo convinti che sia utile arrivare al proibizionismo, perché, avendo raggiunto il gioco d'azzardo volumi notevolissimi, ciò determinerebbe fratture sociali e nuovi spazi di crimine. Riteniamo, invece, utile rafforzare le riforme restrittive, nel segno della tutela della salute dei cittadini e delle comunità. Regioni ed enti locali hanno avviato *iter* legislativi significativi, che a regime prevedranno misure operative e formative: limiti agli orari di apertura delle sale da gioco, distanziometro ovvero il divieto di apertura di sale da gioco e/o servizi commerciali che ospitano *slot machine* entro una distanza, in genere circa 500 metri, da luoghi definiti sensibili, quali scuole, luoghi di culto, ospedali, centri ricreativi e sportivi, luoghi frequentati soprattutto dai soggetti più a rischio, in primo luogo giovani e anziani. Ma questo non basta: c'è bisogno di procedere con un'azione coordinata a livello parlamentare e governativo, per individuare le fasce che distinguono i tipi di gioco per categorie, individuate per persone coinvolte e rischi connessi; formare addetti ai lavori e pubblicizzare il rischio dell'azzardo, studiando nuovi equilibri, che non trasformino il tempo libero di un giocatore in tempo da liberare per consegnarlo ad una ossessione distruttiva. Con lo *stop* imposto dal Covid-19 anche su alcune aree del gioco d'azzardo, cogliamo l'occasione per ripartire in un modo nuovo, che abbia un valore guida assoluto: la protezione di ciascuna persona da catene di sofferenza da cui è difficile e improbabile venire fuori. Mentre alle nuove generazioni chiediamo scusa in nome di un futuro sostenibile, non inchiodiamo i nostri ragazzi in una realtà virtuale fatta di *slot machine* e scommesse, che distraggono da percorsi di vita. Non vi è bene comune nel miraggio della ricchezza costruita su una speculazione. Un agire che non mortifichi i posti di lavoro creati in questo comparto, ma che garantisca che il mercato cui si riferiscono non sia territorio di illegalità e di sofferenza. Vedete, colleghe senatrici e colleghi senatori, ricordo bene i volti fieri degli esercenti di Palermo, quando prima del mio mandato di senatore mi occupavo di contrasto alle ludopatie. esercenti, insieme all'insegna della propria attività, chiedevano di apporre una semplice targa, con scritto: «Un bar senza *slot* ha più spazio per le persone»: semplice, ma nello stesso tempo necessaria di tanto coraggio e fiducia in uno Stato che tutela e garantisce i diritti fondamentali. Se i ragionamenti asettici sui bilanci industriali non dovessero dimostrarlo, è da queste manifestazioni di responsabilità che dobbiamo prendere lezione, monito e spunto per costruire nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle, che nella giustizia sociale ha la sua stella polare, accoglie con favore la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta sul gioco d'azzardo, esprimendo il proprio voto favorevole

Signor Presidente, onorevoli colleghi, «non si arrestano le ondate degli sbarchi dei migranti. Nella notte sono arrivati circa un centinaio di stranieri a bordo di barche di fortuna» ed è questa «solo l'ultima conta, che va ad aggiungersi agli oltre 1.100 migranti che sono sbarcati nel *weekend* sull'isola di Lampedusa, ormai ridotta al collasso». questo è l'inizio di uno dei tanti articoli di giornale, che registrano la situazione, che si ripete ormai da molti anni a questa parte - troppi - sulle nostre coste. Oggi, signor Presidente, non voglio però parlare solo di numeri, che conosce bene anche lei, così come li conoscono bene anche i miei colleghi senatori. Signor Presidente, le chiedo la cortesia di prestare un attimo di attenzione, perché l'argomento è molto importante.

lei, così come li conoscono bene anche i miei colleghi senatori. Oggi vorrei parlare di altro, vorrei parlare di quello che c'è dietro a questi numeri, perché non non basta dire che abbiamo salvato e accolto i naufraghi che i trafficanti di esseri umani mettono in mare, per dire che abbiamo assolto ai nostri doveri umanitari. Non basta e non è sufficiente dire che li abbiamo integrati, solo perché un certo numero di loro è stato collocato in un centro di accoglienza o preso in carico da cooperative e gli abbiamo trovato un lavoro. Non basta, perché dietro ai numeri di questi sbarchi, che noi della Lega contestiamo perché incontrollati *(Applausi)*, ci sono tante vite fragili, tante vite fragili, di cui spesso si perde traccia. Poco più di un mese fa, in Commissione infanzia, ho chiesto conto dei bambini scomparsi

attualmente è stata aggiornata al 30 giugno 2020 e prende in considerazione i bambini scomparsi dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2020. È quindi ovvio che di molti bambini scomparsi non si è saputo più nulla.

Anche se l'Italia rientra tra i Paesi dove scompaiono meno minori rispetto agli altri Stati europei, Presidente, la cosa che mi ha colpito è il fatto che di questi bambini scomparsi il 68 per cento sono minori stranieri, il che significa che su dieci minori scomparsi quasi sette sono stranieri. I dati sui ritrovamenti sono confortanti, per carità, e di questo ringraziamo chi lavora per prevenire e contrastare questo fenomeno. Ma resta sempre una percentuale piuttosto alta di minori di cui non si ha più traccia. Dove finiscono dunque questi minori stranieri? E allora vede, Presidente, a me viene la pelle d'oca quando, in uno dei tanti articoli di giornale, leggo che arrivano sulle nostre coste barconi con centinaia di profughi tra di loro ci sono molte donne, ma soprattutto bambini, la maggior parte senza genitori e - aggiungo io - forse venduti ai trafficanti di esseri umani e che finiranno tra le mani della criminalità organizzata; di loro non si saprà più nulla. Non le sembra, Presidente, che questo sia uno dei tanti motivi per cui è necessario fermare questa disonorevole migrazione incontrollata? La lascio con questa domanda e la ringrazio per l'attenzione.

colleghi, mentre il governo regionale siciliano propone un bando per la progettazione di due termoutilizzatori, in provincia di Enna, in località Dittaino, sta per essere autorizzato un inceneritore. Con un nome roboante ("Piattaforma di recupero risorse idriche tramite essiccazione di fanghi da depurazione e recupero energia termica dalla parte secca"), viene camuffato un inceneritore che brucerà fanghi essiccati, provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue. Sia chiaro: il progetto di cui parlo è complementare alla manifestazione d'interesse per i due termoutilizzatori proposti dal presidente Musumeci. Sarà un terzo impianto che nascerebbe per bruciare fanghi, ma, come si evince dall'elenco dei codici identificativi dei rifiuti (allegato al progetto), sarà autorizzato a bruciare anche altro. La procedura di valutazione ambientale è stata avviata a gennaio 2020, nel silenzio generale, con il benestare delle amministrazioni competenti e nessuna pubblicità dell'atto volta a informare la popolazione; lo stesso Consiglio comunale di Enna non è stato chiamato a esprimersi in merito. L'impianto disterà pochi chilometri in linea d'aria, da alcuni centri dell'ennese come Agira, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Nissoria e Valguarnera: un grande comprensorio agricolo di qualità, dove insistono numerose aziende che trasformano, confezionano e commercializzano prodotti agroalimentari che giungono sulle nostre tavole e all'estero. Questo inceneritore distruggerà materia organica che potrebbe, invece, essere utilizzata per la produzione di biogas e compostata per un successivo utilizzo in agricoltura, se priva di sostanze inquinanti. Mi chiedo quale sia la visione del governo regionale in termini di sviluppo della Sicilia interna, visto che sono 400 i progetti per grandi impianti fotovoltaici già presentati sull'intero territorio regionale, di cui circa 50 in provincia di Enna, che andranno a occupare aree a vocazione agricola. Basti pensare che solo pochi mesi fa erano stati proposti tre siti per lo stoccaggio di amianto, a pochi chilometri da Enna e Caltanissetta, decisione poi revocata. Adesso, come ho denunciato sulla stampa pochi giorni fa, si vuole realizzare un inceneritore nel cuore dell'isola: personalmente, ritengo tutto questo inaccettabile. La volontà della Regione siciliana di bruciare rifiuti è obsoleta, antieconomica, dispendiosa e nociva per l'ambiente e la salute umana. Peraltro, innesca un meccanismo perverso, che farà rallentare la raccolta differenziata, mancando l'obiettivo europeo che punta ad una quota sempre minore di rifiuti da conferire in discarica, uno scenario tragico e antitetico agli indirizzi del *green deal* e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre che del buon senso. Auspico che il Ministero della transizione ecologica faccia chiarezza sulla vicenda e blocchi questa oscura visione del futuro della Sicilia. I rifiuti non si bruciano.

Venezia e la sua laguna siano rimossi dalla prestigiosa lista del Patrimonio dell'umanità è concreto. La decisione finale verrà presa nella prossima riunione del Comitato del Patrimonio mondiale a Fuzhou, in Cina, dal 16 al 31 luglio prossimi, ma nel frattempo Venezia e la sua laguna vengono derubricati nella lista del Patrimonio mondiale e iscritti nella lista dei siti in pericolo. Le ragioni stanno tutte nell'evidente incapacità delle autorità locali e nazionali, che si dovranno prendere la responsabilità di non aver saputo gestire la città e il suo fragilissimo ecosistema, favorendo scelte scellerate opposte ai parametri per i quali Venezia e la laguna sono stati eletti a patrimonio dell'umanità.

chiede fermamente una soluzione di lungo periodo che impedisca l'accesso in laguna alle grandi navi, dirottandole verso luoghi più idonei nelle aree limitrofe. C'è poi il tema dei flussi turistici. L'UNESCO invita infatti Venezia a sviluppare una reale politica di turismo sostenibile, che significa rispettare la città, il suo sistema e, e, soprattutto, i suoi abitanti, danneggiati da altri progetti impattanti che si vogliono fare, come quello che recentemente è stato proposto per collegare Murano alla terraferma, con la distruzione dell'ultima parte di laguna primigenia con altri scali e *terminal* per il turismo di massa. rapporto invita lo Stato italiano a monitorarne da vicino gli impatti della costruzione e del funzionamento e a sviluppare misure adeguate per mitigare eventuali impatti negativi che ci saranno sull'ecosistema della laguna. Quanto a Porto Marghera, la cui presenza di sito industriale altamente inquinato in una delle lagune più fragili del mondo, a ridosso di una città, costituisce da sempre un pericolo ambientale, per cui si chiede finalmente di eliminare progressivamente le attività nel porto di Marghera che hanno effetto dannoso sull'ecosistema. Non poteva passare inosservato anche in laguna Sud il deposito GPL, per il quale si chiede di smantellare l'impianto di stoccaggio In questo elenco è precisato anche che devono essere fermati tutti i progetti di recente presentati per interventi su vasta scala su beni e ambienti rientranti nel sito UNESCO. Soprattutto, pensiamo che si debba bloccare il progetto del collegamento ferroviario a a cappio, a Tessera, che prevede uno scavo di quattro chilometri, profondo 30 metri, a 200 metri dall'acqua della laguna, per la costruzione di un tunnel ferroviario all'interno di un sito tutelato dall'UNESCO stesso, perché quell'area fa parte della Gronda lagunare, che quindi deve essere assolutamente tutelata. Molti altri sono i punti sui quali concordiamo. L'obiettivo dell'UNESCO deve essere la tutela di questo luogo unico, della città e della sua laguna, dei suoi abitanti e della sua identità. Venezia, lo ripeto sempre, non è un'infrastruttura, ma un ambiente complesso e come tale va tutelo perché patrimonio del mondo, come ben chiaramente ha indicato il rapporto UNESCO.